che all'inizio della seduta i senatori Enrico Borghi, Unterberger, Fregolent, Musolino, Paita, Patton, Renzi, Sbrollini, Scalfarotto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

Signor Presidente, intervengo in quest'Aula per denunciare pubblicamente quanto sta avvenendo nelle Commissioni congiunte 1a e 2a.

decine di temi differenti, tutti estremamente delicati. Andiamo da delitti con finalità di terrorismo, modifiche del codice antimafia, revoca della cittadinanza, occupazione di immobili, danneggiamento per manifestazioni, blocchi stradali, detenute madri, accattonaggio, canapa industriale, resistenza a pubblico ufficiale, videocamere per il Corpo di polizia, porto d'armi, informazione per la sicurezza, benefici ai detenuti: un *pot-pourri* di materie, tutte estremamente delicate, che a questa Camera del Parlamento non viene consentito di analizzare ed esaminare in profondità, come esse vorrebbero. Ora, mi si opporrà che i termini sono stati concordati in Ufficio di Presidenza. Ma è pur vero che a più riprese noi abbiamo fatto notare come questo provvedimento sia un disegno di legge che non prevede una scadenza. Non si vede dunque il motivo per cui questa Camera debba essere sottoposta a tale corsa se non per poter sventolare il prima possibile l'ennesima bandierina repressiva che prende di mira soltanto le fasce sociali più deboli. Invece di contrastare e limitare l'emarginazione, in questo modo la si vuole tacitare e sopprimere, come si sta facendo anche con le opposizioni. In Commissione noi abbiamo chiesto lo slittamento quantomeno dei termini per presentare i nostri emendamenti e ribadiamo anche in quest'Aula la richiesta di questa minima tutela delle prerogative delle opposizioni. Si tratta di reale democrazia. Faccio appello, attraverso di lei, allo stesso Presidente del Senato, perché le istituzioni vengano difese nella loro dignità e a noi, come senatori e senatrici, venga consentito di svolgere appieno il nostro lavoro.

Però non posso non sottolineare - come ho già fatto tra l'altro in Commissione - che la mia esperienza di componente della 2a Commissione si modifica molto a seconda di come siamo congiunti.

l'esperienza è straniante, perché pare di appartenere non solo a due Commissioni diverse, ma quasi a due Camere diverse e a due Parlamenti diversi. L'*iter* del disegno di legge sul fine vita,

nelle quali poi ascoltiamo sempre le stesse cose, nel senso che gli auditi rappresentano punti di vista non differenti, ma sempre il medesimo. Per cui noi abbiamo come una sorta di giorno della marmotta, con audizioni che ripetono sé stesse. Si tratta di un disegno di legge che è stato già calendarizzato, perché - ai sensi del Regolamento del Senato - essendo stato presentato da un numero minimo di senatori, avrebbe

non calendarizzato, che ci ha messo sei mesi a essere approvato dalla Camera. Abbiamo dovuto fare una trattativa e - come detto - si è chiuso l'accordo tra i Capigruppo con la decisione di stabilire un numero massimo di audizioni.

molto diverse tra loro. Pensi che noi abbiamo chiesto lo stralcio dell'articolo 31, perché tocca materie delicatissime quanto alla sicurezza nazionale. Si tratta di *intelligence*, si tratta dei Servizi, si tratta quindi di questioni estremamente complicate. Andiamo dalla cannabis *light* all'occupazione delle case; dall'imbrattamento degli immobili alla gestione dei disordini nelle carceri: c'è veramente di tutto e di più.

poi oggi il Presidente, per efficientare i lavori, ci ha detto che, se non intervenivamo, bisognava chiudere la Commissione e cancellare. C'è una pressione

calendarizzato per l'Aula; la Camera da cui esso arriva si è giustamente presa il suo tempo. Veramente non capisco per quale ragione dobbiamo andare a deliberare su un numero così ampio di materie, avendo letteralmente il fiato sul collo e dimenticandoci che si tratta pur sempre di norme penali che incidono sullo *status libertatis* dei nostri concittadini, e quindi, per definizione, andrebbero ragionate e meditate. Non si capisce la ragione della fretta. Mi aggiungo quindi alle preoccupazioni della collega Maiorino, chiedendo a questa Presidenza di

perché quella che è stata fatta dalla senatrice Maiorino e poi dal senatore Scalfarotto è una richiesta che vorrei fosse condivisa anche dai senatori di maggioranza. Guardate, questo disegno di legge

È vero che abbiamo svolto delle audizioni e lo abbiamo fatto con quel criterio che tendenzialmente viene seguito, guardando a un numero di auditi che appaia in astratto ragionevole.

rischia di incidere anche in maniera significativa sulle modalità di azione dei Servizi di sicurezza. Su questo specifico tema

lo voteremo noi senatori. Siamo noi che dobbiamo esercitare un voto in maniera consapevole e, per esercitare un voto in maniera consapevole, dobbiamo avere la possibilità di conoscere e approfondire ciò che stiamo per deliberare. Ho fatto l'esempio dell'articolo 31, ma lo stesso si può fare per tanti altri articoli, tant'è vero che - come abbiamo già più volte segnalato in Commissione - si sta per sta per determinare una prassi molto pericolosa per le prerogative parlamentari, e cioè quella di predisporre dei disegni di legge estremamente eterogenei. Ad esempio, quando audiamo gli esperti, ci accorgiamo che saltiamo da un argomento all'altro. Stiamo contemporaneamente svolgendo le audizioni sul disegno di legge cosiddetto semplificazioni e sul disegno di legge semplificazioni economiche, e quindi sono tre disegni di legge che vanno in parallelo.

Che cosa osta a svolgere un'altra serie di audizioni che ci consenta di colmare quelle parti del disegno di legge che non è stato possibile approfondire, e delle quali sarebbe invece necessario che avessimo tutti quanti la massima contezza? Il rischio è di non essere messi nelle condizioni di poter svolgere adeguatamente le nostre funzioni. far organizzare i lavori delle Commissioni in modo da consentire a ogni senatore di acquisire tutte le informazioni necessarie e gli approfondimenti dovuti e dovuti e da evitare che ci sia la trattazione congiunta di una pluralità di questioni eterogenee, non connesse da alcun rapporto di comunanza con un argomento che, invece, dovrebbe essere ciò che caratterizza ogni disegno di legge. Senatori, trasmetterò al Presidente le vostre richieste.

Il provvedimento, quindi, è già in discussione da oltre un mese. Sono state svolte oltre 30 audizioni e sono stati acquisiti tantissimi contributi scritti da parte di esperti, che sono stati messi a disposizione di tutti i colleghi sulla pagina della Commissione. Attualmente è in corso la discussione generale, con oltre 30 iscritti a parlare.

è stato deciso dalle due Commissioni riunite all'unanimità. Ci sono i verbali e potete andare a controllare. Comprendo le ragioni sostanziali per le quali si chiede di approfondire di più. È chiaro che non si finisce mai di approfondire. Tuttavia, Presidente, mi permetta di farle presente che una richiesta di ulteriori audizioni andava forse formulata in Commissione, prima che in Aula. In Commissione non è mai stata formulata una richiesta di proroga dei termini per la presentazione degli emendamenti. È vero che oggi la senatrice Lopreiato ha formulato questa richiesta intervenendo sull'ordine dei lavori. Ma è anche vero che io ho risposto che, trattandosi di una decisione che riguardava sia la Presidenza della 1ª Commissione, che quella della 2ª Commissione, mi riservavo di confrontarmi con la presidente Bongiorno prima di dare una risposta. Per carità, capisco i toni e la necessità di alzare sempre lo scontro su qualsiasi argomento, ma mi pare che, da un punto di vista procedurale,

Concludo, signora Presidente, chiedendo scusa ai colleghi dell'opposizione, dicendo che ho scordato a casa la museruola.

recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria***

prevede la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Purtroppo, il fenomeno delle aggressioni al personale e alle strutture sanitarie è in tragico e continuo aumento. Secondo un'indagine pubblicata pochi giorni fa dal «Sole 24 Ore», prendendo come riferimento il periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto di quest'anno, non c'è stato un solo giorno in cui un medico o un infermiere, cento dei casi una donna, signora Presidente, non abbia subito una violenza fisica, nella maggior parte dei casi da un paziente o da un parente di quest'ultimo. Al primo posto - guardando al luogo dove si consumano le aggressioni - ci sono i pronti soccorso, al secondo gli interventi degli operatori del 118, al terzo i reparti di psichiatria. La violenza contro gli operatori sanitari è inaccettabile e deve essere contrastata con il massimo del vigore. Non ha solo un impatto negativo sul benessere psicofisico del personale sanitario, ma influisce anche sulla sua motivazione al lavoro; questa violenza compromette la qualità delle cure e mette a rischio l'offerta sanitaria. Tanti medici - l'esperienza quotidiana ce lo dimostra - hanno deciso di abbandonare i pronti soccorso e altri di andare a lavorare nel settore privato, lasciando il settore pubblico, proprio perché spaventati dalle aggressioni e dalle violenze. Questo fenomeno porta anche a immense perdite finanziarie nel settore sanitario. Il Governo, per cercare di contrastare il fenomeno, ha varato il presente decreto- legge. Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, occorre rammentare che la Commissione ha ritenuto di svolgere per l'istruttoria legislativa un ciclo di audizioni informali, ascoltando magistrati, esperti di diritto penale e processuale penale, nonché rappresentanti degli Ordini dei medici. Nel merito, il disegno di legge di conversione consta di quattro articoli. L'articolo 1, in relazione al quale la Commissione ha approvato una modifica formale alla rubrica (la parola «modifica» all'articolo 635 del codice penale è stata sostituita con «modifiche»), introduce un nuovo comma nell'articolo 635 del codice penale, che disciplina il reato di danneggiamento, con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose ivi esistenti, o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. La disposizione prevede anche un'aggravante speciale (la pena è aumentata fino a un terzo) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite. L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i reati di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 inserisce nel secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza il delitto, disciplinato dal secondo comma del già citato articolo 53-*quater* del codice penale, di lesioni personali, commesso a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, e il delitto di danneggiamento, previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale (lettera a-*quater*), come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, testé illustrato. La lettera *b)* del comma 1 inserisce all'articolo 382 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-*bis*, diretto a consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno delle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria. Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente appunto di procedere all'arresto differito quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. Più precisamente, l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato sulla base di documentazione videofotografica - il testo originario, in relazione al quale la Commissione ha approvato una modifica formale, faceva riferimento a documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, che attesti in modo inequivocabile la realizzazione del fatto. In ogni caso, l'arresto dev'essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione del soggetto e comunque entro il massimo di quarantott'ore dal fatto. prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone che il presente decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2

l'inaccettabile piaga delle violenze sugli operatori sanitari non accenna a diminuire, anzi peggiora, facendo segnare in cinque anni un più 38 per cento. Si tratta ormai di un problema culturale: ogni anno sono oltre 130.000 i lavoratori aggrediti. Pensate che dal 1° al 31 agosto non c'è stato un solo giorno in cui un medico o un infermiere (nell'80 per cento dei casi donna) non abbiano subito una violenza fisica. A fronte di questo, la politica può e deve fare di più. Ormai è un bollettino di guerra quotidiano e le vittime sono i lavoratori della nostra sanità, che sono il fiore all'occhiello del settore per la competenza, l'abnegazione, l'empatia e l'umanità con cui svolgono la loro professione al servizio degli italiani e di tutti coloro che arrivano nel nostro Paese. violenze toccano anche i piccoli centri e le periferie del nostro Paese, già fragili dal punto dal punto di vista dei servizi. «So dove lavori, stai attento»: questo è il titolo di un articolo che, nei giorni scorsi, occupava la prima pagina di un settimanale della provincia di Cuneo, la mia provincia. Nemmeno il cuneese purtroppo è esente dalla piaga delle minacce e delle violenze contro i medici e il personale ospedaliero. Sono tanti gli episodi segnalati dalle associazioni di categoria: solo nell'ospedale «Regina Montis Regalis» di Mondovì, a settembre si sono registrate ben quattro aggressioni, con sedie che volavano, letti spostati e tensione altissima. episodi gravissimi, che hanno spinto il sindacato di infermieri e operatori sanitari a sollecitare provvedimenti. Gli episodi ribadisco che sono gravissimi e si moltiplicano quotidianamente e naturalmente

Occorre lavorare per sensibilizzare le persone, che devono capire che gli operatori sanitari fanno solo il loro dovere e nessuna situazione di emergenza può giustificare tali comportamenti. Chi non lo capisce va punito con pene esemplari, questo provvedimento. I posti di lavoro nei pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nei 118 e in ambienti difficili come i reparti psichiatrici non sono più in luoghi sicuri e di questo dobbiamo farci carico. Si tratta di un male sociale che va debellato quanto prima. Che non ci sia più una via d'uscita, altrimenti perderemo il prezioso personale sanitario.

Ma oggi occorrerebbe rivedere queste indennità alla luce dello *stress* correlato, legato alla violenza e al rischio, oppure prevedere una specifica indennità. Al secondo posto tra le vittime di violenza ci sono gli operatori del 118; al terzo, quelli dei reparti di psichiatria. Tra le cause scatenanti di questa aggressività dilagante, ritengo che una delle più gravi sia la mancanza di personale che si riversa sul cittadino che necessita di cure;

le quali nei prossimi dieci anni servirà il 30 per cento di medici in più per garantire il *turnover* del personale sanitario, perché cesseranno di lavorare oltre 50.000 medici e 24.000 infermieri. Serviranno più di 27.000 medici,

e 6.300 operatori sociosanitari, prevalentemente in aggiunta rispetto alla dotazione attuale. Vi è poi il tema delicato (che verrà affrontato) dell'inserimento delle *bodycam* nei luoghi di lavoro esposti a queste tipologie di rischio; un tema su cui occorre una riflessione alla luce dell'aggravarsi della situazione, perché potrebbero essere uno strumento utile per scoraggiare le violenze.

chi compirà un atto di violenza nei confronti del personale sanitario rischia fino a cinque anni di carcere e chi danneggia le strutture sanitarie, multe fino a 10.000 euro; se i danneggiamenti sono stati commessi da più persone, la pena verrà incrementata. Vengono previsti l'arresto obbligatorio in flagranza, ma anche l'arresto in flagranza differita per aggressioni ai danni del personale e nuove linee guida per la videosorveglianza. perché niente può giustificare reazioni violente che diventano ancora più inaccettabili quando vengono perpetrate nei confronti di chi lavora per curare e assistere gli altri che sono in difficoltà. La prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro in ambito sanitario sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, ma anche dei pazienti e delle persone che usufruiscono dei servizi già in condizioni fragili.

però per tutti coloro che lavorano nel settore sanitario con abnegazione, umanità, passione, con grandi sacrifici personali propri dei loro familiari costretti a passare in secondo piano rispetto alle esigenze della professione, noi dobbiamo fare di più: dobbiamo ricordarci sempre che proteggendo tutti gli operatori sanitari

dal 1° al 31 agosto di questo anno, ogni giorno un medico o un infermiere, nell'80 per cento dei casi una donna, ha subito violenza fisica, prevalentemente da pazienti o familiari. Le aggressioni si verificano principalmente nel pronto soccorso seguite da interventi del 118 e dai reparti di psichiatria. Su questa analisi credo che stiamo concordando tutti. Le azioni e le leggi finora adottate non hanno arginato questo fenomeno, che spinge molti professionisti a cercare opportunità all'estero, oltre a quelle economicamente più gratificanti. I luoghi di lavoro, soprattutto in contesti critici come i pronto soccorso e i reparti psichiatrici, sono diventati insicuri per il personale sanitario e in particolare per le donne. Negli ultimi cinque anni, le aggressioni contro i professionisti sanitari sono spaventosamente aumentate del 38 per cento - questo dato ricorre anche nelle relazioni che abbiamo ascoltato adesso

Fattori come lunghe liste d'attesa, mancanza di dialogo tra sanitari e pazienti e assenza di Forze dell'ordine nei momenti critici sono stati citati come motivi significativi alla base di questo aumento. Un'indagine recente ha evidenziato che il 42 per cento dei professionisti sanitari ha subito almeno un episodio di violenza, con un aumento del 40 per cento degli episodi contro le donne negli ultimi tre anni. Nonostante questo allarmante scenario, il disegno di legge in discussione sembra essere solo un palliativo piuttosto che la soluzione o una soluzione reale al problema; ci troviamo di fronte a una battaglia invisibile, con una preoccupante *escalation* delle aggressioni ed è cruciale non solo riconoscere il problema, ma anche evitare soluzioni semplicistiche. La carenza dei professionisti genera un caos nei pronto soccorso e negli ambulatori, le aggressioni in crescita del 24 per cento sono conseguenza diretta di questo sovraccarico. Il 23 per cento delle violenze è collegato alle lunghe liste di attesa. È fondamentale, quindi, considerare questa situazione non come un mero problema normativo, ma come una necessità collettiva che richiede interventi strutturali e coordinati. La formazione continua del personale sanitario potrebbe essere - ed è - una priorità, a nostro avviso: è inaccettabile inviare i professionisti in contesti di alta pressione senza adeguata preparazione. Ogni operatore deve sentirsi dotato degli strumenti necessari per proteggere la propria sicurezza, così come il benessere dei pazienti che assiste. Dobbiamo quindi investire anche in formazione, non solo per migliorare l'esperienza del paziente, ma anche per garantire la sicurezza degli operatori. Inoltre, va rivista la presenza delle Forze dell'ordine negli ospedali, in particolare negli orari più critici. Un'adeguata strategia di sicurezza è necessaria affinché ogni professionista possa svolgere il proprio lavoro senza timori per la propria incolumità. Un approccio multidisciplinare è quindi essenziale per affrontare la violenza nel settore sanitario, con integrazione di competenze psicologiche e sociali. Potenziare la medicina territoriale è fondamentale per migliorare la comunicazione tra cittadini e istituzioni sanitarie, tutelando la fiducia reciproca. È urgente procedere con l'assunzione di personale sanitario e sociosanitario, perché ogni paziente, come ogni operatore, merita un'assistenza di alta qualità e un ambiente di lavoro sicuro in cui sia rispettata la dignità umana. Riguardo all'organizzazione del pronto soccorso, secondo il decreto ministeriale n. 70 del 2015, ci sono *standard* definiti in base al numero degli abitanti: ad esempio, un pronto soccorso DEA di primo livello serve un bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti. Quello che sto dicendo può sembrare un tecnicismo a molti di voi, ma è la sostanza per la quale oggi ci troviamo ad affrontare il sovraffollamento e forse anche una delle necessità che ci spingono a dare a dare più fondi per aumentare il personale e limitare questo sovraffollamento. Se la popolazione, però, supera i 150.000 abitanti, si dovrà attivare un DEA di secondo livello che offre prestazioni più complesse. Ho presentato ben tre interrogazioni per richiedere la riapertura di un pronto soccorso, che si trova a Boscotrecase, in provincia di Napoli, chiuso da quattro anni. Prima della chiusura, il pronto soccorso gestiva un numero considerevole di accessi annui (60.000) ed era ed è un DEA di primo livello. La sua chiusura ha portato a un sovraffollamento nell'ospedale più vicino di Castellammare di Stabia, dove sono stati segnalati diversi episodi di violenza. Questo è un segnale di allerta che non può più essere ignorato

Il sovraffollamento, causato da un'eccessiva presenza di pazienti, colpisce il normale funzionamento del pronto soccorso e trova le sue cause in fattori di ingresso, come per esempio l'invecchiamento della popolazione (che potrebbe essere ed è un fattore in ingresso di una maggiore popolazione nei confronti del pronto soccorso), ma anche i problemi strutturali interni e difficoltà di uscita, dovuti alla mancanza dei posti letto. Dico questo semplicemente per affrontare il problema in modo più organico rispetto a quello che stiamo affrontando noi oggi e per documentare che un atteggiamento del Governo di inasprimento di una norma non risolverà il problema delle aggressioni.

delle pene. Invito tutti a leggere su «PubMed», un portale liberamente accessibile a tutti, sei studi di letteratura internazionale, che offrono una visione complessiva di cosa significhi attuare delle norme per prevenire questi fenomeni. Nessuna delle conclusioni di questi sei studi prevede un aumento di pena; nessuna.

Gli studi suggeriscono che formazioni teorico-pratiche possono ridurre significativamente gli eventi aggressivi. In sintesi, non basta aumentare le pene per risolvere il problema delle aggressioni degli operatori sanitari. Convinciamoci tutti che non è la strada del panpenalismo a risolvere il problema italiano della carenza di personale e anche delle stesse aggressioni. È necessario un piano di assunzione e un contesto lavorativo dignitoso affinché i pazienti possano ricevere assistenza di alta qualità, un piano concreto e un approccio orientato a garantire non solo la sicurezza degli operatori sanitari, ma anche un'assistenza di qualità per i nostri pazienti, per noi. In conclusione, il disegno di legge attualmente in esame non affronta adeguatamente il problema delle aggressioni. Per noi è vitale un approccio più completo e coordinato per migliorare la sicurezza e il servizio sanitario per tutti gli operatori e gli utenti del sistema. Solo così potremo garantire un'assistenza di qualità e la dignità di tutti coloro coinvolti nel sistema sanitario.

di intendimenti e di percezione dei problemi della nostra comunità; una diversità culturale e, ovviamente, una diversità politica con le opposizioni. Questa assise si è aperta questo pomeriggio con degli interventi che sono andati a criticare un metodo, che avevamo espressamente rappresentato ai nostri elettori come caratteristico di un'alleanza che avrebbe governato questo Paese, il centrodestra, che oggi lo sta egregiamente guidando grazie a una *Premier*, a Ministri, Sottosegretari e parlamentari coraggiosi, che hanno dignitosamente la capacità di metterci la faccia e di non sentirsi in imbarazzo nel momento in cui si intende reprimere un comportamento ritenuto dannoso per la nostra comunità. Una serie di comportamenti che, sin dall'inizio di questa legislatura, abbiamo sempre e comunque inteso reprimere. Si ricorderanno i colleghi dell'opposizione che abbiamo da subito inteso far capire quale sarebbe stato il nostro atteggiamento nei confronti di quei fenomeni cosiddetti *rave*. Da lì è iniziata una linea operativa di questa maggioranza, che certamente non si fermerà di fronte ai comportamenti che purtroppo affliggono questa nostra società in maniera veramente preoccupante. È di poche ore fa la reazione convulsa, veramente illogica, immotivata e folle di due giovani che hanno accoltellato un pubblico ufficiale, un controllore a bordo di un treno, per il semplice fatto di aver chiesto loro i titoli di viaggio. è motivo di orgoglio il fatto che alcune delle norme che oggi trovano sede in testi normativi che ci accingiamo a passare da questa Aula portino la firma dei nostri Ministri e dei nostri parlamentari e che ci siano orgogliosamente dei parlamentari che intendono perfezionare quei testi e non arretrare di un millimetro quelle che sono le esigenze di risposta sociale che dobbiamo dare a persone che evidentemente non hanno ben capito che cosa significhi stare in società, stare in comunità, condividere delle risorse, ringraziare coloro i quali quotidianamente si prodigano per soccorrere, soccorrere, per aiutare, per portarsi in aiuto degli altri. Ebbene, troviamo assolutamente inconcepibile che ci siano dei giovani che addirittura a distruggere le proprie relazioni personali, uccidendo una compagna. Poche ore fa questa maggioranza ha onorato il 4 novembre, ha onorato gli uomini e le donne in divisa e gli eredi di quegli uomini e di quelle donne che cento anni fa hanno concluso un'esperienza militare vittoriosa per questo Paese. Oggi sappiamo bene che l'Occidente e il mondo moderno sperano di poter regolare i loro rapporti evitando l'uso delle armi. Questo, purtroppo, spesso non è possibile, ma nella nostra comunità non pistole e coltelli in mano a giovani, a delinquenti, a persone che si trovano purtroppo negli ospedali a rappresentare il loro stato di difficoltà sociale, psicologico, psichiatrico economico. Per noi questo tipo di condotte non può assolutamente trovare nessun tipo di accordo, accondiscendenza o clemenza.

andiamo ad arricchire un quadro normativo che sarà sicuramente di lezione per qualcuno. Le notizie che arrivano in queste ore non ci possono assolutamente consentire di abbassare la guardia. "Il Resto del Carlino" riporta un fatto di poche ore fa, accaduto a Ferrara: si denuda e picchia i sanitari, tra i quali una donna. Il 2 novembre a Civitavecchia un medico è stato preso a pugni

quotidianamente, ma questa maggioranza non intende piegarsi a nessun tipo di comportamento offensivo o lesivo del diritto di frequentare gli ospedali. Permettetemi di concludere

indicava i requisiti degli ospedali, molto diversi da quelli che sono oggi gli ospedali. In quella legge si indicava come obbligatorio almeno una cucina, una dispensa, una lavanderia, un servizio di assistenza religiosa, una biblioteca, una sala riunioni dei sanitari; quasi un luogo familiare, un luogo di accoglienza, un luogo di serenità e di tranquillità, non un luogo dove andare a sfogare i rancori e le difficoltà che - molti dei nostri cittadini devono comprenderlo - non possono assolutamente derivare dal comportamento dei sanitari, dei funzionari e degli uomini e delle donne che operano nel campo sanitario con delle prestazioni che hanno soltanto lo scopo di salvare le persone. [**Presidenza del Se c'è qualcuno che pensa di poter impunemente utilizzare - perché poi il problema si sposta anche nelle aule giudiziarie - uno strumento giudiziario per condividere le proprie lotte politiche e addirittura dimenticare l'esponenziale rischio a cui espone tutto il Paese nel momento in cui si debbono anche applicare quelle norme, la nostra attività politica evidentemente poi si occuperà anche di rappresentare correttamente al sistema giudiziario quali siano i rischi di interpretazioni. Purtroppo lo abbiamo visto nelle scorse ore, foriere di confondimenti che trascendono in ambito politico. Per quanto

di mettere in pericolo la sicurezza del nostro Paese andando a confondere, nell'esercizio delle loro funzioni, metodi e atteggiamenti che sono prettamente politici e che dovrebbero essere semmai rappresentati correttamente in questa sede, come alcuni colleghi ex magistrati hanno fatto candidandosi e venendo qui a esprimere le loro idee politiche. prima di tutto, a nome del mio Gruppo Italia Viva, voglio esprimere la mia e la nostra solidarietà a tutto il personale sanitario e ausiliario sociosanitario, ai nostri medici, ai nostri infermieri *(Applausi)*, che stanno subendo oramai quotidianamente violenze e aggressioni in quei luoghi che sono deputati alla cura, alla tutela della nostra vita, del nostro stare bene.

c'è la necessità di intervenire condannando sempre ogni forma di violenza (ci mancherebbe). Mi faccio anche un'altra domanda: perché siamo arrivati a questo punto? È doveroso interrogarci su questo come parlamentari. Siamo arrivati al punto che dobbiamo garantire la sicurezza nei luoghi di cui si occupa chi lavora e opera a tutela della salute. Ciò vuol dire che siamo di fronte certamente ad un imbarbarimento della società,

mai giustificare nessun tipo di violenza. Accade, come è stato detto anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, perché è il sistema sanitario che non regge più. Colleghi e colleghe, lo abbiamo visto lo abbiamo visto e ascoltato nelle audizioni in nella 10a Commissione qualche giorno fa, ma anche ieri nella Commissione bilancio. La Fondazione GIMBE, che da sempre ci dà la fotografia reale di quello che succede nel nostro Paese, ci dice che da qui

tutto il lavoro del ministro Schillaci, che più volte ha fatto un appello al suo stesso Governo per avere più risorse economiche a sostegno anzitutto delle assunzioni di medici e infermieri, perché sono

personale socio-sanitario e infermieristico. Nello stesso tempo, abbiamo la necessità di investire nell'assunzione di più personale sanitario, in stipendi più alti e sicuramente in una maggiore formazione e dignità del personale medico. Ricordo che queste persone sono state i nostri angeli ed eroi durante il periodo del Covid. Li abbiamo ringraziati e detto loro che il sistema sanitario sarebbe cambiato, che avremmo investito di più

lavoro. È chiaro ed evidente che non serve e non si può solo pensare di militarizzare i luoghi della salute.

anche negli ospedali e nei luoghi della salute. Tuttavia, non si può pensare di avere soltanto questo

mi auguro - e voglio ancora sperare - che il Governo possa pensare seriamente a come lavorare per una sanità più equa e giusta su tutto il territorio nazionale. Infatti continuiamo ad assistere a un abbandono continuo, da parte dei medici e degli infermieri, dei nostri ospedali, per non parlare delle strutture di emergenza (pronto soccorso) e altri luoghi, proprio per i motivi che ho appena elencato. Allora io dico: siamo ormai alla vigilia di una finanziaria e nelle audizioni di ieri anche Confindustria, che ha sempre un atteggiamento molto attento anche nei confronti di chi governa, ha detto che così non si può andare avanti. È una manovra finanziaria senza una visione, è una manovra finanziaria dove si va a colpire ancora una volta il ceto medio manovra finanziaria che ancora una volta indebolisce politiche sociali di *welfare* che sono alla base di un sistema, anche culturale ed educativo, che deve cambiare nel nostro Paese. nel nostro Paese. Se si continuano a tagliare risorse nella scuola, nella sanità e nelle politiche sociali, cosa ci possiamo aspettare? Una società migliore, o una società che diventa più aggressiva e più violenta, dove il disagio, a cominciare da quello giovanile, è un disagio che facciamo finta di non vedere ogni giorno? Allora, quando parliamo di politiche attente ad una società migliore, anche questo provvedimento doveva diventare l'occasione per investire in un sistema di *welfare* e per dare risposte con politiche

su cui cresce una società, non l'imbarbarimento di cui stiamo parlando ogni giorno con provvedimenti che vedono l'introduzione di nuovi reati o l'inasprimento delle pene. Ma è mai possibile che non pensiamo che dovremmo investire nell'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri figli, delle nostre comunità? La ciliegina sulla torta è arrivata ieri ma avrò occasione di parlarne anche in altri interventi - con il taglio netto e violento sui nostri Comuni, attraverso una manovra finanziaria che va a tagliare sulla sanità, sul sociale, sulle politiche del territorio, sul dissesto idrogeologico e sulla sicurezza, nonostante quello che stiamo vivendo anche in queste settimane con il maltempo. Per tutte queste ragioni - lo dico con grande rammarico - avremmo preferito chiaramente esprimere un voto favorevole a questo provvedimento, ma - come dirà bene il mio collega Scalfarotto nella dichiarazione di voto - ci dovremo astenere, perché ancora una volta avete perso un'occasione per costruire un provvedimento serio a partire dalle politiche culturali e sociali di cui ha tanto bisogno il nostro Paese.

tutto il Senato dovrebbe ringraziare i medici, soprattutto quelli che si adoperano per salvare la vita e sono sicuramente tanti i casi di buona sanità nei pronto soccorso. Li dovremmo ringraziare per tutte quelle persone che giornalmente i pronto soccorso dei nostri ospedali riescono a

Dobbiamo dire però che il problema va affrontato logicamente anche con altri atti normativi a 360 gradi, perché evidentemente la mancanza di medicina territoriale in molte Regioni e in molte situazioni crea anche un accesso anomalo: spesso infatti le strutture dei pronto soccorso sono intasate perché c'è un accesso anomalo di codici che non hanno la caratteristica di urgenza;

proprio in questi mesi sta facendo sopralluoghi in tutti gli ospedali italiani, per parlare con i medici, che logicamente ci chiedono una mano. I concorsi per i pronto soccorso però stanno andando deserti, quindi non è che non ci siano: la verità è che il personale e i dottori non vogliono più lavorare nei pronto soccorso, perché

assieme su un tema che ci accomuna. Vediamo anche dalla discussione che si sta svolgendo in Aula che il tema ci accomuna, perché il decreto-legge in esame è in continuità con il lavoro fatto nella scorsa

personale sanitario. Eppure, ancora una volta, questa maggioranza ha chiuso a qualsiasi possibilità di confronto, bocciando tutti gli emendamenti dell'opposizione, anche se non erano previsti costi. Non mi riferisco solo agli emendamenti che chiedevano di stanziare più risorse o di strutturare meglio il territorio, ma anche a tutto quel pacchetto importante di emendamenti che chiedevano alla maggioranza di lavorare sulla prevenzione. Addirittura è stato bocciato un emendamento che chiedeva l'obbligo di esporre nei pronto soccorso, nei luoghi in cui più facilmente avvengono aggressioni, dei cartelli informativi per dire ai cittadini che esiste questa legge e che se si aggredisce personale

per i direttori generali della valutazione dei rischi, per responsabilizzare sempre di più la dirigenza sanitaria; sono state bocciate le proposte di inserire più videosorveglianza. Insomma, è stato bocciato tutto e questo è il motivo per cui noi ci asterremo, perché riteniamo che invece questa normativa poteva e doveva essere fatta meglio. Di cosa parliamo quando parliamo di aggressione al personale sanitario? Non desidero ripetere ciò che i colleghi hanno già detto, ma è evidente che siamo davanti a una vera e propria emergenza sociale, sociale, a un fenomeno preoccupante, che io speravo si fosse fermato in pandemia, quando abbiamo chiamato eroi quegli operatori sanitari *(Applausi)*. Gli operatori sanitari che oggi vengono aggrediti sono gli stessi che erano chiusi negli scafandri durante il Covid, sono gli stessi che portavano sul viso i lividi delle mascherine; quegli eroi oggi invece vengono di nuovo aggrediti. aggrediti. È un fenomeno preoccupante e ce lo raccontano i numeri di quell'osservatorio a cui faceva riferimento anche il senatore Trevisi, che è stato inserito sempre in quella famosa legge Grillo. Signora Presidente, prima di quella legge, si stimavano circa 2.000 aggressioni all'anno; oggi sappiamo che i numeri sono quasi dieci volte più alti e si parla di 18.000 aggressioni all'anno. Questo perché molte di quelle aggressioni non venivano denunciate dal personale sanitario. Oggi, invece, c'è l'obbligo della procedibilità d'ufficio anche grazie a quella legge. Come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, il 40 per cento degli operatori sanitari, durante la propria carriera, subisce un'aggressione. Le aggressioni colpiscono le donne nell'80 per cento dei casi e colpiscono soprattutto gli operatori che lavorano negli ospedali del Sud Italia e in particolare nei reparti di pronto soccorso, nell'emergenza urgenza territoriale - quindi il 118 -, nei reparti di psichiatria, carceri, di cui finora non si è parlato. Le cause, come abbiamo visto anche da uno studio pubblicato recentemente, sono legate perlopiù alla carenza di personale, alle liste d'attesa lunghissime, alla mancanza di comunicazione, ma io dico che in generale la causa è legata alla fragilità che sta vivendo in questo momento il nostro Servizio sanitario nazionale a causa dei tagli che sono stati operati dal 2008 al 2018 e a causa della cattiva programmazione e spesso della cattiva gestione della sanità. Dobbiamo dire - non lo facciamo troppo spesso in quest'Aula - che non ci si può improvvisare a gestire la sanità dopo, per esempio, aver semplicemente fatto poche ore di un corso regionale. Serve una legge seria, che finalmente sleghi le nomine dei vertici della sanità dalla politica. *(Applausi)*. Abbiamo presentato anche in questa legislatura una legge, la n. 187, che chiede proprio di inserire dei criteri meritocratici per i direttori generali, per i direttori sanitari, per i direttori amministrativi. Faccio un appello alla maggioranza:

che i bravi medici, le nostre eccellenze restino in questo Paese, perché si sentono valorizzate. *(Applausi)*. Facciamo gestire la sanità a chi ha tutti i titoli per farlo, inseriamo anche dei criteri più stringenti di valutazione, per esempio, dell'operato dei direttori generali, valutando anche la riduzione del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, così come la riduzione delle liste d'attesa. Oggi spesso nessuno di questi criteri viene considerato considerato nella valutazione dell'operato di un direttore generale. Le politiche sanitarie portate avanti in questi anni, come diceva anche il collega Mazzella, hanno fatto sì che venissero smantellate quelle reti territoriali che invece erano un filtro potentissimo, proprio per evitare il sovraffollamento dei grandi ospedali. dei pronto soccorso che devono gestire dei numeri veramente incredibili, ho personalmente accompagnato dall'allora ministro Speranza venti medici del pronto soccorso del Cardarelli che avevano consegnato la lettera di dimissioni al Ministro perché si rifiutavano di lavorare in quella condizione. Abbiamo dei reparti di osservazione intensiva breve, che sono dei reparti adiacenti al pronto soccorso in cui le persone dovrebbero stare per poche ore e che sono diventati dei reparti di degenza, come, ad esempio, nel caso del Cardarelli. Abbiamo una medicina territoriale gestita unicamente dai medici di medicina generale, che non riescono più a fare da filtro. Anche questa riforma si dovrà fare e dobbiamo cominciare a parlarne in quest'Aula,

che possa evitare il sovraffollamento degli ospedali. Eppure, anche quei soldi l'attuale maggioranza non riesce a spenderli, se dei fondi PNRR ad oggi è stato speso circa il 10-12 per cento, quindi molto al di sotto della soglia prevista. C'è un grande lavoro culturale da fare, questo l'hanno detto in tanti e io lo condivido, perché bisogna fare in modo che i cittadini ritrovino quella fiducia nelle istituzioni, che significa anche fiducia nel personale sanitario che ci ha in cura, ma c'è soprattutto un grandissimo lavoro strutturale da fare e non serve solo incrementare i presìdi di polizia, che in quest'ultimo anno sono aumentati moltissimo, eppure sono aumentate anche moltissimo le aggressioni, quindi non è quella la ricetta. La ricetta per ridurre le aggressioni, così come per ridurre le liste d'attesa, passa attraverso due canali: il primo è l'assunzione di personale sanitario e il secondo è la creazione di un filtro agli ospedali che parta dal territorio. poi soprattutto investire risorse. Colleghi, non c'è bisogno della calcolatrice per capire che in questa legge di bilancio ci sono a stento le risorse che serviranno per la gestione ordinaria della sanità e non si potrà invece assumere il personale sanitario che serve. Voglio concludere, Presidente, ricordando a tutti - e questo lo faccio da medico - che quando un medico si laurea presta un giuramento, il famoso Giuramento di Ippocrate, in cui giura giura innanzitutto di non nuocere alla salute delle persone che assiste. E, allora, vorrei veramente che anche i cittadini di questo Paese facessero un giuramento, che è quello di non aggredire chi è lì solo per prestare aiuto e soccorso perché questo, a mio avviso, è il fondamento su cui si deve basare un Paese che si definisca civile.

mi sia consentito di approfittare della discussione generale per portarvi un mio punto di vista. Pur non essendo una acerrima sostenitrice dell'introduzione di nuovi reati o dell'inasprimento delle pene, quanto piuttosto della necessità di farle rispettare ed applicare, per queste fattispecie si tratta di estremi rimedi, poiché è del tutto evidente infatti che bisogna fermare l'ondata di violenza nei pronto soccorso, negli studi medici, nelle corsie degli ospedali, nelle strutture per anziani e disabili, fino ad arrivare alla tutela dell'incolumità dei professionisti nei servizi veterinari, ma anche sui treni. Precondizione del benessere organizzativo e della serenità degli operatori in attività così essenziali per tutti noi è infatti l'assenza di violenza sui luoghi di lavoro ed è per questo che dobbiamo provarle tutte anche sul piano penale, altrimenti ci verremo a trovare per colpa di pochi senza sanità e senza assistenza, senza controlli e senza prevenzione, per mancanza di operatori, perché uno che al mattino esce di casa, sia pure motivato da grandi ideali, non può pensare di tornare a casa la sera, tumefatto o accoltellato. È apprezzabile che in parallelo si stia intervenendo per togliere ogni pretesto soprattutto di tipo emotivo, andando a incidere sui tempi di presa in carico nei pronto soccorso e sulle liste d'attesa, sulle misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, agendo in estrema sintesi, sulle cuspidi delle criticità nei tempi di risposta ai bisogni e per traguardare livelli di appropriato intervento sanitario ed assistenziale, territoriale, specialistico ed ospedaliero. È per questo che puntiamo sull'accelerazione degli *iter* normativi che abbiamo promosso per il riordino dell'emergenza urgenza, per l'evoluzione delle specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie e sociosanitarie, nonché per l'effettivo potenziamento della medicina territoriale in prevenzione ed assistenza primaria, andando a far confluire i peculiari contenuti del processo di revisione e di riorganizzazione promosso nel disegno di legge governativo n. 1241 e nei due collegati ordinamentali alla legge di bilancio all'uopo dedicati, in sinergia con quanto previsto dal Governo e in una strategia complessiva di universalità e di sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale, secondo principi di responsabilità e di etica solidale, individuale, professionale e collettiva in tutta la filiera, filiera, con nuove regole di ingaggio dei prescrittori e degli erogatori, indispensabili per marginalizzare tutte le inappropriatezze, gli sprechi e le disfunzioni e per finalizzare adeguatamente le risorse, limitate ma non scarse. Risorse che quindi debbono essere orientate per lo sviluppo delle risposte delle risposte appropriate alle necessità di sistema, investendo per dare di più, pur costando di meno, ed educando che per rivendicare i diritti bisogna ricordarsi i doveri, non esistono diritti a costo zero, *c'est-à-dire* che ognuno di noi deve anche pagare le tasse, per quanto può per davvero, perché anche nella giungla non c'è un pasto gratis. Vi ringrazio. Signora Presidente, colleghe e colleghi, stiamo discutendo in questo momento di un decreto-legge che riguarda la sicurezza del personale sanitario, mentre è in corso nel nostro Paese lo sciopero generale dei lavoratori delle ferrovie (di tutte le compagnie delle ferrovie) esattamente per un tema analogo, cioè per l'aggressione che è avvenuta a Genova nei giorni scorsi. Credo che sarebbe utile

come un luogo attraverso il quale scaricare rabbia, rancori, difficoltà di comprensione, forme di disagio e anche forme di aggressione criminale. Questo non è normale. I numeri li hanno già dati i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto. Non è normale un tale livello di aggressioni e di aggressività rispetto ad un personale che normalmente ha come attività fondamentale quella di rispondere alle esigenze dei cittadini e di dare loro dei servizi. Credo che non si possa liquidare un tema di questo tipo semplicemente pensando che aggravare le pene e introdurre nuove fattispecie di reato di per sé determini un clima differente da quello in cui siamo.

perché anche in quei giorni eravamo di fronte a un episodio drammatico avvenuto in un pronto soccorso. Tale emendamento diceva che era possibile prolungare, attraverso l'esame dei filmati e delle videoregistrazioni, la flagranza di reato. Se era solo questo l'obiettivo, ho una domanda: perché non lo si è fatto lì e abbiamo dovuto respingere quell'emendamento in quell'occasione per fare un decreto-legge che alla fine dice solo questa cosa? Credo che davvero questo sia un modo, da un lato, di svilire il Parlamento e il lavoro che tutti e tutte noi facciamo quotidianamente, ma anche, dall'altro lato, un'idea di costruire un messaggio politico secondo il quale si può rispondere alle questioni di questo Paese solo attraverso l'istituzione dei reati e delle pene. e delle pene. Non credo che questo sia un messaggio utile e lo dico con grande sincerità; non credo che aver aggravato le pene impedisca questo tipo di aggressioni. Penso invece che abbiamo due domande da farci; possiamo magari dare delle risposte diverse, ma proviamo a porci queste domande. Molte colleghe e colleghi hanno parlato della necessità di un grande lavoro culturale: sono assolutamente d'accordo, ma spesso si parla di grande lavoro culturale senza che ciò si traduca in una decisione su quali siano i temi rispetto ai quali tale lavoro è necessario. Ve lo dico dal versante di chi ha continuato in questi anni ad occuparsi di lavoro: possiamo fare una riflessione su quanto abbiamo svalorizzato il lavoro pubblico su quanto abbiamo gettato la croce sul fatto che, poiché non funzionavano i servizi e non c'era una giusta responsabilità, erano i lavoratori pubblici a non rispondere alle esigenze dei cittadini, e non il sistema che non investiva più risorse e che non assumeva da vent'anni della pubblica amministrazione? Se continuiamo a dire che sono i lavoratori a non rispondere alle esigenze, noi gli abbiamo messo un bersaglio in fronte. Possiamo domandarci perché, in un Paese come il nostro, nel giro di due anni il personale medico e sanitario è passato da eroe ad sanitario è passato da eroe ad aggredito in qualunque occasione? Non è successo qualcosa che riguarda anche il nostro modo di parlare di questo tema? Sono scandalizzata: il Senato ha ospitato, nel giro di un mese e mezzo, due riunioni che erano un grande abbraccio ai no-vax e a chi fa quotidianamente un lavoro di messa in mora e in discussione di quanto ha fatto la sanità in questo Paese. I toni che abbiamo usato nella discussione rispetto alla Commissione Covid di nuovo portano lì, cioè all'idea che c'è un mondo che è colpevole, quello della sanità, che ha reagito

un clima di diffidenza verso i lavoratori pubblici e, dall'altro, un clima di diffidenza verso la medicina e l'attività scientifica. Possiamo mettere tutte le pene che volete, tutti i presìdi di polizia che volete *(Applausi)*, ma quei lavoratori li lasciamo esposti giorno dopo giorno al fatto di essere vissuti come colpevoli. colpevoli. Capisco che è una bella scorciatoia: tutte le volte ci raccontate che possiamo creare un nuovo reato, inasprire le pene, aggiungere cinque aggravanti e così via. Poi c'è la frase classica di tutti i vostri decreti,

mentre poteva essere esattamente l'occasione per provare a discutere di cosa non funziona nel Servizio sanitario nazionale e come gli operatori del Servizio sanitario nazionale sono assolutamente lasciati da soli ad affrontare ogni emergenza. ogni emergenza. Aggiungo che invalgono sempre di più nel Servizio sanitario, ma in generale nei servizi pubblici, delle cose che chiunque abbia un po' di attenzione a come sono i luoghi di lavoro si domanda se funzionino. Pensiamo davvero che ci possano essere dei lavoratori che lavorano in luoghi aperti al pubblico, al servizio pubblico, e che possono essere da soli e che non si pensi che quella condizione di solitudine diventa anche una condizione che li espone a qualunque reazione, a qualunque disagio, a qualunque difficoltà? Un tempo era dato per scontato che nelle situazioni di tensione e di difficoltà non si potevano mai lasciare dei lavoratori da soli; men che meno si potevano lasciare da soli lavoratori che non sono attrezzati a gestire situazioni di difficoltà di questo tipo. Saper fare il buon medico o il buon infermiere non vuol dire essere anche in grado di gestire una situazione di disagio, di violenza o di difficoltà. Forse bisognerebbe pensare a come li formiamo. Forse bisognerebbe investire delle risorse perché ci sia una capacità, che riguarda tutto il personale di quei luoghi, che abbia delle reazioni. Investire in formazione dovrebbe essere sempre il primo dei pensieri

I pronto soccorso non possono continuare a essere l'unico luogo a cui tante, troppe persone si rivolgono per avere una risposta di salute. Costruiamo noi stessi l'emergenza se non diamo una risposta a tutto questo. questo per significare che non è che vada male in sé. Anzi, i medici e gli infermieri che abbiamo audito hanno apprezzato che ci fosse questa norma. Non abbiamo alcun dubbio che ci sia una volontà e una disponibilità ad avere almeno questa come parafulmine sui temi della sicurezza. Qualunque risposta a chi si sente esposto viene ovviamente presa positivamente. Non possiamo però immaginare che il nostro ruolo si limiti a questo.

Credo che dobbiamo smetterla di perdere le occasioni e pensare che grandi questioni come la sicurezza del nostro personale sanitario possano diventare solo una bandierina. Dovrebbero invece diventare un intenso cantiere per ridare al Servizio sanitario nazionale quella funzione che ha sempre avuto e che, forse, ci aiuterebbe anche a diminuire un malessere sociale diffuso che non fa mai bene a una società.

Sono quotidiane le aggressioni verbali e fisiche ai danni di medici, infermieri e personale sanitario, che sono gli stessi uomini e donne che durante la pandemia abbiamo chiamato eroi. Le notizie che emergono all'onore delle cronache sono quelle più gravi e drammatiche e rappresentano appena la punta dell'*iceberg* di una situazione preoccupante e diffusa che crea un clima di paura sul posto di lavoro per chi opera nel campo della salute. La relazione al Parlamento dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie mostra come nel 2023 siano state oltre 16.000 le segnalazioni di episodi di aggressione, con violenza fisica o verbale, minacce o contro la proprietà. Nei due terzi dei casi le vittime sono state professioniste donne. La professione più colpita è quella degli infermieri, che il più delle volte sono coloro che si trovano in prima linea, a contatto più ravvicinato con l'utenza. I luoghi più a rischio sono risultati essere i pronto soccorso, le aree di degenza e le strutture di salute mentale. Nei dipartimenti di emergenza sono soprattutto i parenti ad aggredire il personale, dove le lunghe attese spesso slatentizzano rabbia e frustrazioni represse. Qui il sovraffollamento e la carenza di posti letto e di personale contribuiscono a istigare comportamenti aggressivi; il medico e l'infermiere vengono visti non più come coloro che si prendono cura, ma come coloro che colpevolmente trascurano i pazienti e i loro familiari. Altro luogo a rischio sono i reparti di psichiatria, dove è il paziente ad aggredire in condizioni di acuzie psicopatologica o in una condizione di intossicazione da sostanze. Non c'è da stupirsi se, dopo la pandemia, le aggressioni siano in aumento, tanto che un recente sondaggio mostra come l'81 per cento degli operatori sanitari riferisce di essere stato vittima di aggressioni fisiche o verbali. Il dato ancora più allarmante è però che ben il 69 per cento dei sanitari non denuncia l'aggressore. Si tratta di un fenomeno non solo nazionale. Infatti, guardando al contesto europeo e mondiale, si osserva come in Europa si è assistito a un incremento delle aggressioni del 36 per cento negli ultimi cinque anni, in linea con quanto accade nel resto del mondo. Il Governo è già intervenuto con il decreto-legge n. 34 del 2023, che rafforza il sistema normativo penale, aumentando le pene per chi aggredisce operatori sanitari e rafforzando la presenza di presìdi fissi di polizia presso le strutture dotate di dipartimenti di emergenza, poi con il decreto legislativo del marzo 2024, dove si è prevista la procedibilità d'ufficio indipendentemente dalle denunce della persona offesa. Ora, con il decreto-legge in discussione, si adotta finalmente l'estensione dell'arresto in flagranza differita anche alle violenze operate nei confronti dei professionisti sanitari. Com'è noto, l'arresto in flagranza differita dà la possibilità al personale di pubblica sicurezza di arrestare entro le 48 ore il soggetto che ha procurato violenza e quindi assicurarlo alla giustizia. Si tratta di uno strumento molto utile, già adottato in contesti quali le manifestazioni sportive o i reati inerenti alla violenza domestica. Quelli del Governo sono provvedimenti importanti, che evidenziano la strategia che il Governo e il ministro Schillaci in particolare stanno portando avanti per il contrasto a questo odioso fenomeno che ha raggiunto livelli ormai intollerabili. Oltre alle misure legislative è però necessario affiancare un lavoro che guardi un cambiamento culturale e una profonda riflessione sulle cause che sono alla base del fenomeno della violenza ai danni del personale sanitario e, più in generale, sul ruolo che medici, infermieri e personale tutto hanno nella società e su come la percezione di queste figure si sia evoluta nel corso del tempo. Nel corso del dibattito da più parti è stato sottolineato come il nostro Servizio sanitario nazionale stia attraversando un periodo di grave crisi e le aggressioni rappresentano solo il più drammatico epifenomeno della situazione. Le ragioni sono molteplici e vanno ricercate certamente nel definanziamento subìto dal sistema sanitario nazionale con tagli dal 2010 al 2019 di 37 miliardi e con la chiusura di 125 ospedali nel periodo dal 2011 al 2021, ma è innegabile come questo Governo stia cercando di invertire la rotta con stanziamenti da record previsti per il 2025 in 136,5 miliardi e per il 2026 in 140,6 miliardi Altra causa va certamente ricercata nella carenza di personale sanitario, legata ad una programmazione per troppi anni inadeguata *(Applausi)*, con la conseguente carenza di personale. Spesso assistiamo a concorsi pubblici per medici e infermieri che vanno deserti e si è costretti a ricorrere a gettonisti o a personale straniero per consentire il funzionamento dei reparti, specie nell'emergenza-urgenza. Ma vi sono molte altre ragioni, altrettanto importanti, di tipo culturale ed organizzativo, che contribuiscono alla crisi del nostro sistema sanitario nazionale e che meritano di essere analizzate perché non estranee al cortocircuito che sfocia nel fenomeno delle aggressioni. Chi vi parla, per la propria storia professionale di oltre trent'anni di servizio come medico in strutture ospedaliere pubbliche e per una storia familiare di cinque generazioni di medici, educato in una visione della professione come missione di assistenza e cura al malato, vuole stimolare una riflessione su come il ruolo del personale sanitario e del medico in particolare sia percepito nella società. È finita l'epoca nel quale la parola del medico non veniva in alcun modo messa in discussione. Oggi il rapporto medico-paziente si è completamente trasformato e non di rado il medico si trova a dover convincere il paziente dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle sue prescrizioni: un cambio epocale che sta compromettendo il mutuo rapporto fiduciario, indispensabile perché vi sia una corretta alleanza terapeutica fra medico e paziente. Una condizione dovuta certamente ai grandi progressi della medicina, alle ultra specializzazioni, al consumismo terapeutico, ma soprattutto all'informazione spesso distorta che il paziente riceve ed elabora sulle capacità che la scienza possa curare tutto e subito. I mezzi di informazione sono pieni di notizie di malasanità e poco spazio rimane per la tanta buona sanità che ogni giorno viene erogata con dedizione, passione e professionalità da medici e infermieri, spesso tra mille difficoltà organizzative. Abbiamo assistito negli ultimi vent'anni, spesso nel silenzio della politica, ad una crescita esponenziale dei contenziosi legali per responsabilità professionale in ambito sanitario, contenziosi che contribuiscono a intasare i nostri tribunali, aumentando i costi assicurativi e nel 95 per cento dei casi si risolvono in un nulla di fatto, favoriti da chi specula su pazienti e medici, la cui conseguenza più evidente è stato il fenomeno della medicina difensiva che da qualche decennio sta logorando il nostro sistema sanitario e le nostre finanze, con conseguenze che ricadono in primo luogo sui pazienti, a cui vengono prescritti accertamenti spesso inutili, costosi e talvolta anche invasivi, aggravando così le liste di attesa della sanità pubblica. Quello a cui assistiamo, colleghi, è un pericoloso cortocircuito, in cui sia medici che pazienti stanno perdendo la fiducia l'uno nell'altro, il medico non riesce a svolgere la professione in serenità, nel timore di essere denunciato o aggredito, e il paziente teme di essere oggetto di un ennesimo episodio di malasanità. È in queste dinamiche che si collocano gli episodi di aggressione: bisogna sforzarsi allora di costruire una nuova cultura della cura e una sana relazione tra medico e paziente, in cui si ritrovino empatia e umanità, in un'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia, sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando anche quello della comunicazione come tempo di cura. Va riscoperta la deontologia medica e occorre far sentire ai pazienti che il medico è il loro miglior alleato, che mette a disposizione la sua professionalità sempre per il loro bene, e che qualsiasi atto di violenza commesso contro di lui è commesso contro se stessi. Allo stesso tempo, occorre ridare dignità alle professioni sanitarie: istituzioni, associazioni di pazienti e *mass media* devono dare tutti il proprio contributo perché si ritrovino il rispetto e la giusta considerazione per coloro che hanno dedicato la propria vita alla cura degli altri. Solo così si potrà ridare orgoglio agli operatori sanitari per riscoprire le vere e migliori motivazioni che li hanno portati ad abbracciare la professione. È necessario un processo culturale, che faccia comprendere la complessità che caratterizza la relazione medico-paziente e corregga l'idea che responsabilità corrisponda a colpa e che la medicina possa dare sempre a tutti risposte miracolistiche. C'è una grossa differenza nella pratica clinica fra insuccesso ed errore: il primo si chiama complicanza, un evento possibile in ogni azione umana, che in medicina e chirurgia è correlato al grado di complessità dell'atto medico, nel quale rientrano i limiti oggettivi delle conoscenze scientifiche e la singolarità dei malati e dei contesti in cui si opera. Oggi, purtroppo, l'insuccesso troppe volte viene scambiato per errore e colpa, intasando i tribunali e rovinando ingiustamente la vita professionale di molti. I giovani medici si allontanano dalle specialità più a rischio e scelgono di andare a lavorare all'estero, in un processo favorito da speculazione e malafede, tanto da incrinare quest'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia. Per superare le violenze e il conflitto fra cittadino e personale sanitario bisogna che insuccesso ed errore vengano definiti in modo chiaro,

In conclusione, colleghi, questo provvedimento rappresenta un tassello importante del lavoro che il Governo sta portando avanti per rilanciare il nostro sistema sanitario, un importante contributo per restituire la giusta serenità agli operatori sanitari, ma molto rimane da fare, perché, oltre a questi necessari interventi, occorre uno sforzo ancora maggiore sul piano culturale per sensibilizzare i cittadini e rinsaldare il rapporto di fiducia tra pazienti e professionisti sanitari.

dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.100, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.101, 2.0.13, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7.

Signora Presidente, nella discussione generale abbiamo parlato pochissimo di diritto e moltissimo di sanità, di salute. Il Governo ci ha mandato il Sottosegretario di Stato per la giustizia perché si tratta di norme penali. Tuttavia, come fa questo Governo, la norma penale è una scusa

dei risarcimenti, che aspettino; nel frattempo mandiamo Delmastro Delle Vedove a Palazzo Madama e si farà un po' di cultura in sanità.

loro fanno il piano carcerario, ma i numeri dei carcerati aumentano talmente tanto che il loro piano carcerario andrà sempre aggiornato ai nuovi numeri. Insomma, noi stiamo cercando di suggerire di provare, per esempio, a usare le sanzioni amministrative, perché esistono. Dato che anche in questo caso stiamo andando a normare nuovamente condotte che sono già illecite, perché il reato di danneggiamento da quel dì è previsto dal codice penale, io dico di lasciar stare questi reati che esistono: li abbiamo avuti per tanto tempo e non sarà il vostro nuovo reato o la vostra nuova pena a fermare

sottolineare il fatto che si tratti di un reato commesso contro beni destinati alla cura delle persone, stabiliamo una bella sanzione amministrativa anche importante facciamo in modo che venga applicata con una cartella esattoriale, senza mettere in moto un processo penale con tutto ciò che ne deriva. Tra l'altro, la sanzione è anche immediata, come ci ha anche detto in audizione il rappresentante dell'ordine dei medici: quando gli ho chiesto se, secondo

si capisce più di diritto di certi esperti del diritto che scrivono cose di questo genere. Anche prendendo ispirazione dall'ordine dei medici, abbiamo provato a farvi vedere come si può fare una norma che va a incidere su un comportamento indesiderato, sbagliato e illecito, ma senza tirar sempre per i capelli il codice penale, il processo penale e anche la galera, perché non se ne può più. più. Imparate. Vi abbiamo scritto un emendamentino molto grazioso, che potrete applicare anche i prossimi sciacallaggi e ai prossimi reati che riuscirete a inventarvi, dimostrate anche una creatività - devo dire - fuori dal comune: uno non direbbe mai che le destre sono così creative, eppure ogni volta ci stupite con nuove norme. Io lascio qui anche a futura memoria una specie di emendamento *omnibus:* lo approviamo oggi e ce lo teniamo buono anche per i prossimi esercizi di creatività del nostro Governo *law and order*, legge e ordine.

abbiamo rilevato un impegno delle Forze di polizia per creare dei punti di presenza che in molti casi già c'erano, mentre in altri casi sono stati rafforzati negli ultimi anni e dotati di telecamere. Ovviamente il personale deve pensare a tante esigenze, ma ci sono dei punti fissi, anche con la presenza di telecamere, che possono poi attivare, in casi di emergenza, ulteriori interventi delle strutture di zona. Tuttavia, in molti ospedali, soprattutto nelle grandi città, c'è anche personale di istituti di vigilanza privata che è contrattualizzato, ingaggiato dalle aziende ospedaliere, che contribuisce, negli accessi, negli ingressi negli ospedali, nelle zone limitrofe al pronto soccorso, a un'attività di vigilanza, come accade del resto nei Ministeri, nelle banche, negli aeroporti e in tanti altri luoghi. Noi siamo ben consapevoli dell'apporto fondamentale degli istituti di vigilanza che, regolati dalla legge, svolgono un'attività di concorso e di sostegno, sgravando - pensiamo al controllo bagagli negli aeroporti o a tante altre funzioni - le Forze di polizia da un lavoro impegnativo, ma che può essere svolto da forze concorrenti.

perché anche nelle discoteche c'è un addetto all'ingresso, ma non è questo l'esempio, si tratta di figure *extra* legge. Per le attività degli istituti di vigilanza regolate dalla legge, autorizzate dalla prefettura, contrattualmente ingaggiate dalle aziende ospedaliere, riteniamo che si dovesse estendere questa tutela, cioè l'aggravante prevista nel caso una persona aggredisca un poliziotto, un infermiere o un medico: anche nel caso ad essere aggredita sia una persona di un istituto di vigilanza, oltre alle responsabilità penali già esistenti, scattano queste aggravanti. una piccola lacuna che abbiamo voluto colmare; dopo un confronto con il Governo si è arrivati a una riformulazione, ma il principio credo che allarghi le tutele e le sanzioni. Volevo sottolineare questo aspetto perché credo che tutti i colleghi possano condividere lo spirito e la sostanza dell'emendamento

per quanto riguarda l'emendamento 1.7, del senatore Giorgis, che l'ha presentato in qualità di Presidente del Comitato per la legislazione. Non è un parere contrario nel merito, ma essendo stato

«a valutare l'opportunità di», compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

quindi, questi fenomeni molto deprecati debbano coinvolgere, oltre che personale sanitario, infermieri, medici, o esponenti delle Forze di polizia, anche il personale delle strutture di vigilanza privata, esso sia tutelato da questa garanzia rafforzata, proprio per sottolinearne il contributo alla sicurezza e al controllo dell'attività degli ospedali e la funzione complementare - come dice l'emendamento - di queste realtà. L'emendamento 1.500 colma quindi una piccola laguna. Ringrazio anche il Governo per la collaborazione e la riformulazione a cui siamo arrivati.

ho sperato che risolvesse uno dei grandi misteri di questo decreto-legge. Nella mia dichiarazione di voto tornerò poi sul tema delle sanzioni penali per decreto-legge. Questo decreto-legge stabilisce che il danneggiamento, e quindi la reclusione da uno a cinque anni - non è che stiamo scherzando stiamo scherzando - si applica alla persona che abbia distrutto, disperso, deteriorato o abbia reso in tutto o in parte inservibili cose ivi esistenti nell'ospedale o

per il solo fatto che esiste lì dentro, ti becchi cinque anni di galera. Io lascio l'ombrello nella sala d'attesa, il mio ombrello esiste, qualcuno distrugge l'ombrello che esiste nell'ospedale e si becca cinque anni di galera. Non so se adesso uno vuole interpretare - vedo il collega Delrio, per il quale nutro grande stima - ma qua c'è scritto così. Io mi pongo il problema del giudice. mi pongo il problema del giudice. Oggi in Commissione affari costituzionali siamo stati invitati a leggere il *dossier* del Senato. Peccato che poi i magistrati, quando applicano la legge, non leggono il *dossier*, ma leggono la norma che noi approviamo qua stasera.

schifezza, non mi viene altro termine. Invece purtroppo non è così e quindi, in dichiarazione di voto, annuncio il voto contrario del mio Gruppo, perché, se non andiamo a risolvere quel problema, qualsiasi altra cosa non serve.

sanare alcune delle cose più evidentemente sbagliate di questa norma. Tuttavia, questo emendamento accoglie una serie di osservazioni che noi stessi avevamo fatto e che avevamo messo in appositi emendamenti, quali però - secondo una prassi abbastanza consueta della maggioranza - sono stati trasformati in emendamenti della maggioranza, non riconoscendo il lavoro che viene fatto dall'opposizione. Per cui noi ci asterremo, anche se riconosciamo che sono piccoli miglioramenti dell'attuale norma, così come noi avevamo richiesto in Commissione.

è molto colto e sa bene qual è la normativa attualmente vigente. Una fattispecie del genere sarebbe scriminata con la speciale tenuità del fatto e, quindi, nessun giudice agirebbe

per dire che voteremo a favore di questi emendamenti perché vanno a risolvere un problema, perché sopprimono le parole «ivi esistenti o comunque», e quindi si lascia che siano destinati all'uso sanitario. Mi lasci però anche dire una cosa, per il suo tramite, signora Presidente. mi si dica che si possono introdurre un reato e una pena su una fattispecie assurda, perché tanto c'è l'attenuante della speciale tenuità del fatto, indica in modo molto chiaro come si legifera in materia penale in questa Camera. Intanto io metto il reato, poi eventualmente ti appelli all'attenuante. Ma, se ho fatto una cosa che non ha alcuna offensività, in uno Stato di diritto non diventa un reato perché lo Stato di diritto è fatto sulla base del principio che tutto ciò che non è vietato è lecito. *(Applausi)*. Altrimenti noi rovesciamo questo paradigma e ci troviamo, senza accorgercene, in un posto che assomiglia pochissimo a quello disegnato dalla nostra Carta costituzionale. Questo ragionamento - e non mi va per niente di scherzare in questo caso - veramente non lo posso accettare, signora Presidente.

dove non si usa il diritto penale senza tener conto del peso che la norma penale importa dentro l'ordinamento giuridico e nella vita delle persone.

strumento reso possibile dalle moderne tecnologie, che però va utilizzato con grande grande attenzione e in modo molto restrittivo. Noi stiamo discutendo un disegno di legge delega sull'intelligenza artificiale. Se cominciamo a dire che, grazie alle tecnologie, possiamo diventare

però, perché su quella strada uno comincia a mettere delle bellissime telecamerine con riconoscimento facciale ad ogni angolo e vi vi garantisco che la repressione del crimine diventa un gioco da ragazzi a quel punto, perché "come te movi te fulmino", come si dice a Parigi. Il problema è che noi ci mettiamo a utilizzare sempre più spesso questo metodo, perché adesso lo facciamo per questa fattispecie, ma è una cosa che questo Governo comincia a fare e a dire: grazie alla videoconferenza o alla telecamera, io ti arresto in flagranza, anche se non sei in flagranza. Allora, presento questo emendamento soppressivo per dire alt,

lo ringrazio per questo e aderisco alla sua battaglia e nello spirito con questo emendamento. Vi dico attenzione, e non perché il reato sia meno grave. C'è tutta l'attenzione l'attenzione a quello che succede, se c'è un'aggressione al personale medico o paramedico. Ma, quando cominci a fare l'eccezione, poi dove disegni la linea, dove tracci il confine diventa difficile e il confine si sposta sempre di un po'. Per questo noi voteremo favorevolmente a questo emendamento.

poi far sì che il personale sanitario sia comunque pronto ad affrontare determinate situazioni. Non è semplice: nel momento in cui parliamo di un numero contenuto di medici o di personale come infermieri, come si fa a gestire una situazione che già chiaramente si verifica in un momento di urgenza, perché vuol dire che si sta agendo per curare e intervenire su una persona e

le persone (medici, paramedici, psicologi e psichiatri) che si occupano della salvaguardia della nostra salute vengono messe in crisi per la loro salute. Signora Presidente, io sono un esperto: il mio bisnonno, un ginecologo, nella sua clinica sbagliò tutto su di me e nacqui con una notevole disabilità, che, devo dire, mi ha permesso, nonostante tutto, di esprimermi, per qualcuno anche troppo. Stasera, parlando con l'amico medico del Senato Federico Marini, ci chiedevamo com'è possibile che ci sia stata un'inversione di tendenza. Signora Presidente, io non sono d'accordo né sugli allarmismi, né sulla

cultura. Qui si fa politica e la politica la si fa sui punti scomodi, critici, se vogliamo dolorosi, perfino sugli atti di violenza contro persone che ci sostengono. negli ultimi anni c'è stata una delegittimazione dell'apparato complessivo; ci sono stati provvedimenti, soprattutto da parte dei Governi tecnici, di impoverimento numerico del personale che hanno creato solitudine di ruoli e difficoltà nell'ottemperare a tutte le loro funzioni. Nonostante tutto, non è solo questo. Abbiamo avuto l'enfatizzazione di farmaci miracolosi e di

spunti negativi, ma diciamocela tutta: questo provvedimento non risolve, ma è d'aiuto per questo personale che si porta dietro il carico di dolore, poiché non solo si cura con difficoltà, ma si torna a casa con l'angoscia del giorno dopo. A mio avviso questo provvedimento intanto in parte risolve e dà certezze, ma soprattutto fa sentire meno solo il personale messo in crisi.

Abbiamo avuto il coraggio di far politica su un punto così difficile. Signora Presidente, dica ai colleghi da parte mia che mi occupo da oltre mezzo secolo

problemi di nicchia. Sapete qual è il problema più grosso di queste persone con malattie rare, con problemi spesso insolubili ed insoluti? È la solitudine. *(Applausi)*. È la solitudine che noi dobbiamo colmare - certo - dando un riferimento economico maggiore, ricominciando a sbloccare il *turnover*, ci mancherebbe altro, e questo si farà, anche se in un momento così critico a livello economico, ma

nel breve periodo. Credo che davvero vadano ammirati un Governo e dei parlamentari del Senato e della Camera che sostengono un provvedimento in un momento così difficile, su un tema così difficile come ricostruire la fiducia fra medico e paziente, che non può essere impaziente, perché la fretta è davvero sempre cattiva, pessima consigliera. Dobbiamo, questo sì, con i mezzi di comunicazione di massa che parlino di questo provvedimento, dare due garanzie: che chi ferisce la psiche o il corpo di una persona che ci difende, al di là di tutto, commette un reato grave, sempre perché tra l'altro rompe la cosa più importante, la fiducia del medico o del paramedico in sé stesso. Quante volte sono stato minacciato nel servizio di salute mentale da persone con difficoltà, per un *raptus* del momento? Ma intanto ho sempre lavorato in *équipe* e poi non mi sono mai sentito solo rispetto a chi mi aiutava a livello legale e amministrativo.

noi dobbiamo essere dalla parte di chi difende la salute delle persone, soprattutto nei punti critici come i pronto soccorso, il 118, i servizi psichiatrici che in questo momento, dopo il Covid, hanno enormi difficoltà nella gestione della salute mentale. Dobbiamo dare un segnale fortissimo schierandoci dalla parte di chi sta nel giusto amministrando con eroismo la nostra salute. Non possiamo essere mai dalla parte di chi rompe, anche a livello psicologico, anzi soprattutto a livello psicologico, la tranquillità di chi gestisce la cosa più delicata e di maggior valore della nostra società, la salute nostra e soprattutto dei nostri cari. Ho Ho ascoltato con molta attenzione, certamente, soprattutto chi difende tranquillamente, lealmente, intelligentemente questo prodotto legislativo, ma ho ascoltato, come sempre, con tanta attenzione l'opposizione e non si offendano i colleghi che stimo molto,

che promuove e difende un provvedimento così coraggioso, così complesso da portare avanti una sfida di

orgoglio di appartenenza la propria disabilità cui faccio riferimento molto di rado, e dire con questo orgoglio che sono orgoglioso di questo provvedimento, al di là di tutto. Auguri a tutti.

la produzione di norme penali non conosce sosta nella XIX legislatura. Ci incontriamo continuamente per tirare fuori norme penali. E quindi mi tocca, essendo l'unico rappresentante del mio Gruppo in quella Commissione, illustrare alcune questioni che non sono proprie soltanto di questo provvedimento, ma che sono diventate una sorta di *fil rouge*, dando anche un segno del modo di legiferare di questa maggioranza.

con un'idea che ovviamente contrasta in pieno con quella che ci era stata illustrata anche dal ministro della giustizia Nordio quando il Governo, ormai più di due anni fa, entrò in carica. Ricordo distintamente quell'audizione; il Ministro ci raccontò di un diritto penale minimo, di un uso della norma penale risicatissimo, impiegato soltanto quando proprio indispensabile. Ci ricordò del valore della presunzione di innocenza e del diritto alla riservatezza. Tutte cose molto belle, ma in realtà, come sappiamo, questa è la legislatura che passerà alla storia per aver introdotto norme penali anche a tutela dell'orso marsicano. *(Applausi)*. Non voglio infierire, ma se questo è il diritto penale minimo, ci siamo completamente sbagliati. sbagliati. È una questione di fondo basilare perché ha anche a che vedere con il rapporto fiduciario con questa Camera. Io ho sentito dire delle cose, ho quindi espresso il mio voto di fiducia, in quel caso contrario, ma i colleghi della maggioranza hanno espresso il voto di fiducia a favore del Governo su un programma che non è quello che il ministro Nordio e il suo Ministero stanno portando avanti. Questo è il contrario di quello che Nordio ha detto che avrebbe fatto. Viene da dire ai colleghi della maggioranza che se quel voto di fiducia l'hanno espresso su quel programma, oggi dovrebbero votare con noi contro questi provvedimenti.

decreto-legge *rave*. Questo nuovo Governo, finalmente un Governo politico, con una grande maggioranza politica con una grande visione, riunisce il Consiglio dei ministri per la prima volta e che fa? Un decreto-legge sui *rave* per introdurre una norma penale. Ci siamo già detti molte volte, ma io non mi stancherò, signora Presidente, fino alla fine della legislatura, di dire che le norme penali non si fanno con i decreti-legge. Sappiamo che non c'è un divieto assoluto,

Per definizione, quindi, quella norma non avrà un'immediata applicazione, perché tu oggi stabilisci la norma, ma la norma sarà applicata più avanti. Allora uno dice: sì, ma io creo l'effetto deterrente. Qui però va detta una cosa: attenzione, perché la norma penale, con tutta la sua deterrenza, va ragionata. Bisogna pensarci, bisogna approfondire; le norme penali incidono sullo *status libertatis*, cioè sulla libertà dei nostri concittadini. E, quando noi mettiamo mano alla legge per limitare la libertà dei nostri concittadini, dobbiamo fare le norme come si deve; dobbiamo ragionarle, dobbiamo fare in modo che siano equilibrate, dobbiamo fare in modo che siano scritte bene, dobbiamo fare in modo, per esempio, di confrontarci con gli studiosi. Noi facciamo audizioni, lo dico anche a beneficio della scolaresca che ci osserva; quando noi legiferiamo, invitiamo degli esperti cattedratici che ci consigliano e ci spiegano se ci sono complessità sistematiche e se ci sono difficoltà applicative. Invece come viene approvato un decreto-legge? Si riunisce il Governo, si chiudono in una stanza a Palazzo Chigi 20-22 persone, quanti sono i Ministri di quel Governo, si riaprono le porte e quella norma è già viva nell'ordinamento giuridico. Quindi, senza aver fatto alcuna consultazione, alcuna riflessione e alcun pensiero, il Governo si riunisce, finisce la riunione e quella norma esiste. Poi c'è un altro problema: se la norma già esiste, deve essere scritta bene, perché noi sappiamo che quel decreto-legge vive per sessanta giorni, fintantoché viene convertito in legge. E cosa accade ogni volta, signora Presidente? La stessa maggioranza, spesso il relatore, ci portano emendamenti al decreto-legge in fase di conversione. Per spiegare sempre ai non tecnici del diritto, accade il decreto-legge, come approvato, è entrato in vigore così com'era; ma, dopo soli due mesi, c'è una nuova norma penale modificata da chi l'ha scritta. Quindi chi l'ha scritta ci sta dicendo: lo so che l'ho scritta male, perché, se non l'avessi scritta male, non la modificherei. Quindi abbiamo una seconda norma penale e queste due norme si succedono nel tempo in modo così vicino da creare enormi problemi applicativi. Quante volte da questi scranni abbiamo detto: se vi rendete conto, quando scrivete i decreti-legge, che li scrivete male, per carità smettetela smettetela di fare norme penali per decreto-legge, perché poi, come anche in questo decreto-legge, presentate emendamenti per modificare il decreto che avete già posto in essere. Questo non va bene, è una pessima abitudine che va eradicata. Non se ne può più. Non so veramente come dirlo.

quello stesso bene privo di valore intrinseco e magari anche economico diventa un bene giuridico tutelato con la sanzione della reclusione fino a cinque anni. Perdonatemi, colleghi, non si può legiferare così.

anche in questo caso vi siete inventati, e chissà quante altre volte andrete ad applicarlo, questo concetto della flagranza differita. Utilizzo l'ultimo minuto di tempo a che noi, nonostante si tratti di un provvedimento di legge insufficiente, carente e inguardabile, alla fine ci asterremo perché capiamo le buone intenzioni e perché, anche se, come è noto, di buone intenzioni sono lastricate le vie per l'inferno (come anche in questo caso), si vuole tentare di dare un messaggio alla sanità e agli operatori della sanità.

pagati; fatelo proteggendo la scienza: da quei banchi quanto abbiamo sentito proteggere i no-vax anche con provvedimenti di legge? *(Applausi)*. Questo fa male ai medici molto di più. Non è che riparerete il danno che fate alla scienza e gli operatori della sanità con questo decreto-legge. Allora, la mia accorata preghiera è di smettere di utilizzare le norme penali come delle foglie di fico per coprire le vergogne e di cominciare a fare le cose concretamente. Se questo era un atto di attenzione nei confronti della sanità pubblica, prendete un altro provvedimento che si chiama legge di bilancio e metteteci i soldi. Questa roba invece serve a tutto tranne che a dare un segnale alla sanità pubblica. Tuttavia, proprio perché si tratta di una buona intenzione di un qualche genere, ci

incominciamo a dire le cose molto chiaramente. Questo Governo ha un'idea "manettaria" delle problematiche e pensa di risolverle introducendo nuovi reati, pene più severe, maggiore carcerazione e via dicendo.

picchia le porte e via dicendo. Il problema è affrontare questa drammatica situazione. Come si fa ad affrontare il problema

Poi la maggioranza può decidere, come ho detto più volte, perché io non voglio assolutamente mischiarmi con la maggioranza, però vivaddio ci saranno pure delle esperienze e delle proposte che l'opposizione avanza che abbiano un senso. Invece no;

risolviamo le questioni di questo Paese. Per questa ragione ritengo anch'io che sia stata un'occasione persa. Proprio perché il problema c'è, anche noi ci asterremo, però il dato vero è che questa è un'occasione persa, perché non si è voluto affrontare nel modo in cui va affrontato un tema che è drammatico. Offrite una soluzione che non cambierà neanche una virgola della

non posso non partire da un disagio, perché, come tutti voi, non avrei mai immaginato di dover intervenire e dover trattare un decreto-legge contro la violenza sul personale sanitario. che fino a poco tempo fa almeno io ritenevo non immaginabile, da nessun punto di vista. Purtroppo, quella quasi riverenza del passato nei confronti di chi si curava di te e dei tuoi cari è stata sostituita da un'indifferenza e addirittura un'ostilità: un qualcosa che - ripeto - io non avrei mai immaginato, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà. è quello che sta accadendo. Dovremmo ripristinare se non questa buona riverenza, almeno un rispetto e una gratitudine verso chi si occupa dei nostri mali, della nostra salute e del nostro corpo. Purtroppo, però, fino a che tutto ciò non verrà ripristinato, dobbiamo occuparci di creare nuove situazioni giuridiche che possano tutelare il personale sanitario e la nostra comunità, i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie. Questo decreto-legge - ringrazio il relatore Zanettin, perché ha ben seguito il provvedimento, per come ci ha illustrato i contenuti in quest'Aula all'inizio della seduta - rappresenta una risposta concreta a un problema che purtroppo si sta verificando in modo diffuso nel nostro Paese. Garantire la sicurezza di chi si occupa della nostra salute - siamo tutti d'accordo - è fondamentale per assicurare quelle condizioni di tranquillità e di vivibilità di cui le nostre strutture ospedaliere hanno necessità assoluta, anche per non spaventare chi volesse intraprendere questa carriera e rischia oggi di non guardare a quel pronto soccorso in particolare, ma non solo, che è in un certo senso il primo impatto e l'eccellenza della cura al bisogno immediato della persona e che viene vista invece con una trincea dalla quale quasi fuggire.

non può mai giustificarsi, in questo caso ancora di più, e non possiamo assolutamente affrontare con indifferenza tutto ciò che sta accadendo. Le pene previste sono importanti, perché quando si parla di reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10.000 euro, stiamo parlando di pene che ci auguriamo tutti possano introdurre una vera deterrenza, anche se facciamo fatica a pensare che questa sia davvero una soluzione a un problema come questo. Non credo sarà sufficiente e tantomeno non è piacevole né condivisibile addirittura

modo, danneggiare le strutture, i macchinari e i presìdi medici è un fatto odioso e non accettabile, perché non è solo una violenza verso chi lavora e chi utilizza questi strumenti, ma verso tutta la nostra comunità, verso tutti noi e verso le nostre risorse che lì vengono impiegate. ritengo giusto - e ringrazio il relatore Zanettin, che l'ha spiegato bene, ma poi chi non vuol capire non capisce - quando si parla di beni esistenti anche nelle pertinenze di una struttura ospedaliera, voler tutelare quelli del personale sanitario (come l'auto altri beni che possono essere individuati e colpiti da chi purtroppo, ormai l'abbiamo visto, con una furia insensata, può pensare di prendersela non solo con la persona, ma anche con le cose della persona). Dopodiché,

il suo richiamo, perché effettivamente stiamo assistendo a cose che hanno poco senso rispetto alla realtà e alle sue interpretazioni. Il tema Il tema innovativo più importante che viene introdotto è certamente che, per assicurare i responsabili alla giustizia, si introduce appunto la possibilità dell'arresto in flagranza. giusta la previsione dell'arresto in flagranza, come lo è perfino quella della flagranza differita per i reati commessi nei confronti di professionisti sanitari che sono lì a tutelare la salute nostra e quella dei nostri cari e delle nostre comunità. quindi opportune le modifiche agli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale: si tratta di interventi puntuali

far sapere che il legislatore ha deciso di stabilire pene così importanti, perché si tratta di reati gravi, che, lo ribadisco, colpiscono non solo gli operatori sanitari, ma tutta la comunità che ruota attorno a loro, quindi tutti noi

per dare le risposte che i cittadini si aspettano e che quindi è doveroso dare. questo decreto-legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, sociosanitario, ausiliario e di assistenza e cura, nonché del danneggiamento di beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria. Purtroppo, a malincuore, signor Presidente, devo dire che ci siamo astenuti in Commissione. In considerazione del tema trattato, che interessa allo stesso modo maggioranza e opposizione, poteva essere il classico provvedimento approvato all'unanimità;

Il fenomeno delle aggressioni contro il personale sanitario, sociosanitario e di assistenza è un problema crescente e allarmante, che mina la sicurezza di chi è impegnato a garantire cure e supporto alla cittadinanza. Atti di violenza fisica e verbale, nonché danni a beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria stanno aumentando a ritmi preoccupanti. Questi eventi non solo compromettono la salute e la serenità degli operatori, ma intaccano anche la qualità dei servizi e la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario. Nelle ultime settimane un drammatico episodio di violenza si è verificato al Policlinico di Foggia (purtroppo più eventi si sono verificati a Foggia), dove circa 50 persone hanno fatto irruzione nel reparto di chirurgia chirurgia toracica in segno di protesta per la morte di un familiare durante un intervento chirurgico. Il personale sanitario si è visto costretto a barricarsi in uno stanzino per sfuggire alle aggressioni, subendo danni fisici e psicologici evidenti. Io non so se avete visto le immagini che sono girate molto sia sui TG che sui *social*. Una dottoressa è rimasta addirittura ferita ad una mano e un chirurgo è stato colpito al volto durante l'assalto, mentre si attendeva l'intervento delle Forze dell'ordine per riportare la calma. Questi avvenimenti, signora Presidente, evidenziano una situazione di emergenza che richiede una risposta rapida ed efficace per garantire la sicurezza dei lavoratori sanitari, sempre più esposti a episodi di violenza, anche da parte di chi dovrebbe riporre in loro fiducia e rispetto.

sono presto detti e, come sempre, riguardano il merito del provvedimento, come abbiamo detto anche durante l'illustrazione degli emendamenti. Il testo originario proposto racchiudeva delle problematiche di natura tecnica, che sono state prontamente evidenziate dalla parte politica

e comunque lo faremo presente anche durante l'esame del citato provvedimento. Noi, attentissimi, abbiamo quindi evidenziato questo problema, che non ha natura assolutamente politica, ma espressamente tecnica

quale noi proponevamo una deroga per i reati del codice rosso; come al solito, io ho urlato l'importanza di questo emendamento sia in Commissione che in Aula,

ai principi che puntualmente evidenzio in sede di Commissione, cioè il rispetto del principio di uguaglianza oltre a quello della tassatività, della determinatezza della norma penale, con giusto e adeguato bilanciamento tra le pene. le pene. Siamo intervenuti con un'attività emendativa ispirata a tali principi, dove si è voluto precisare il perimetro di applicazione della normativa, indicando i luoghi esclusivamente di emergenza ed urgenza, considerando anche i mezzi di soccorso e indicando, in caso di danneggiamento, solo ed esclusivamente quei beni mobili ed immobili ivi esistenti o comunque destinati al servizio sanitario. Signora Presidente, secondo lei questo è stato sufficiente? No, non è assolutamente sufficiente. Se parliamo di un reato, parliamo di una condotta delittuosa, come già ho precisato al momento dell'illustrazione degli emendamenti, parliamo di una fattispecie delittuosa già posta in essere, già consumata, parliamo quindi di un accanimento sulle pene, con un intervento sempre più afflittivo, ma cosa si fa per la prevenzione? Assolutamente nulla, tant'è che i nostri emendamenti sono stati dichiarati improponibili. Avevamo previsto il registro mancati infortuni su cui annotare le segnalazioni sulla

di un emendamento molto simile del senatore Potenti; tutto va benissimo, ma quello che diciamo noi del MoVimento 5 Stelle non va mai bene. Abbiamo previsto presìdi di Polizia di Stato o sistemi di videosorveglianza, cartelli informativi (lo abbiamo precisato anche in sede di illustrazione degli emendamenti), campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione per il personale finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto. Inoltre, abbiamo precisato l'esigenza di interventi *post* reato, abbiamo quindi previsto il congedo per le vittime di aggressione, nonché

che consiste nel garantire il diritto universale alla difesa e all'accesso alla giustizia, principi fondamentali per ogni democrazia. Un sistema di gratuito patrocinio senza limiti di reddito può inoltre essere decisivo per tutelare i diritti delle vittime di violenza e per consentire l'accesso alla giustizia nelle cause di rilevante interesse pubblico o costituzionale. Questa misura garantirebbe dunque equità e parità di accesso alla giustizia, permettendo a tutti di usufruire di una difesa adeguata e libera da vincoli economici. Tutto questo chiaramente reclama investimenti nella sanità che oggi risulta, ahimè, abbandonata. La sanità pubblica italiana versa in uno stato preoccupante, preoccupante, caratterizzato da carenze strutturali, scarsità di risorse e investimenti insufficienti che stanno compromettendo la qualità e l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini. A fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione e di una domanda di assistenza sanitaria in continuo aumento, dell'obsolescenza delle infrastrutture e della mancanza di attrezzature moderne, di fatto quello di fatto quello che stanziate per la sanità anche in questo disegno di legge di bilancio si rivela assolutamente inadeguato e insufficiente. Questa situazione si riflette in liste d'attesa sempre più lunghe, che costringono molti cittadini a ricorrere al settore privato, creando di fatto una disuguaglianza di accesso alla cura basata sulle disponibilità economiche e purtroppo questo voi lo sapete bene, si investe pochissimo nella sanità pubblica e si propende purtroppo molto per la sanità privata, chiaramente in disprezzo verso coloro che non riescono ad affrontare le spese, come se il diritto alla salute fosse solo per i ricchi e non per i poveri. Anche il personale sanitario è in sofferenza, la carenza cronica di medici e infermieri porta a condizioni di lavoro difficili e spesso insostenibili, con turni massacranti che mettono a rischio il benessere degli operatori e la qualità delle cure. È evidente che senza un piano di investimenti seri e strutturali, la sanità pubblica non sarà in grado di sostenere le sfide future, lasciando una parte crescente della popolazione senza assistenza adeguata e minando il diritto alla salute, alla salute, come dicevo poc'anzi, e nulla cambierà con la prossima finanziaria. Presidente, colleghi e colleghe, il provvedimento sarebbe stato meritevole di essere votato all'unanimità se solo fosse

Poco posso aggiungere a quanto già hanno espresso i miei colleghi in discussione generale; la senatrice Cantù e il senatore Bergesio hanno approfondito in particolare i temi riguardanti la condizione stessa della vita dei sanitari, che diventa

anni, arrivando quasi a porre in dubbio quello che fino a vent'anni fa era un fondamento del nostro stesso vivere sociale e della nostra società.

Nell'attesa di questa ardua sentenza, non possiamo noi, come Governo e maggioranza di centrodestra, non dare una risposta a questa richiesta costante di poter avere una società in cui si possa liberamente vivere. Si vive liberamente nel momento in cui si rispettano le regole. Uno dei primi principi che dobbiamo avere è il rispetto del lavoro. Stiamo parlando in particolare della professione sanitaria,

Sarebbe forse banale ricordare le notizie apparse quotidianamente sui giornali che raccontano di fatti, anche tragici, che hanno colpito il personale medico nell'esercizio della loro attività.

Di certo il contesto in cui stanno operando i sanitari, soprattutto all'interno delle strutture ospedaliere, è particolarmente delicato e grave. Vi sono questioni che riguardano il carico di lavoro, la retribuzione, la responsabilità civile verso terzi, organici, tematiche che questo Governo sta affrontando una ad una per sopperire a vuoti

sanitari. Non possiamo limitarci, come vorrebbe fare qualche parte della politica, semplicemente a scandalizzarci e ad indignarci. Non basta dire che sono degli eroi per rendere una professione esercitabile o appetibile per le nuove generazioni. Dobbiamo dare delle risposte e questo decreto-legge dà delle risposte che si uniscono a quelle già adottate in altri provvedimenti che ora non ricorderò,

è una previsione sul reato di danneggiamento. Stiamo parlando di danneggiamento e di chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, distrugge

aiutando la singola persona che ci lavora, ma stiamo aiutando un intero sistema, nel quale noi stessi viviamo

attuale. Le polemiche e le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Noi vogliamo agire sui temi, come abbiamo sempre fatto come Gruppo Lega, in modo serio e profondamente pragmatico.

1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni

ci siano risorse, misure di prevenzione e misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità di rispondere alle esigenze delle persone. Invece se si apre il provvedimento si scopre che questo provvedimento (misure di contrasto alla violenza) si compone solo di due articoli, che recano il primo

Ora, cari colleghi, il punto di questo decreto-legge è esattamente questo: voi titolate misure di contrasto alla violenza e al danneggiamento e poi fate un provvedimento che non porterà alcun risultato per raggiungere quell'obiettivo. *(Applausi)*. Non porterà alcun risultato perché sapete meglio di me che aumentare le pene non serve ad impedire i fenomeni e le condotte. Non è quella la strada, l'avete già provato in mille altre circostanze. È la strada più facile, perché è quella che consente di dire all'opinione pubblica che noi stiamo affrontando il fenomeno, noi stiamo correndo ai ripari, ed è a costo zero,

per affrontare un problema così complesso, così rilevante e così importante. Ha ragione la mia collega Susanna Camusso, che vi ha fatto un elenco delle cose che servono. È un problema di natura culturale; è un problema di risorse; è un problema di atteggiamento nei confronti della sanità pubblica: di questo bisogna occuparsi se si vuole affrontare in maniera seria un problema di questo genere, e non facendo l'ennesimo provvedimento bandiera e manifesto, che non servirà a nulla. servirà a nulla. Lo dico ai nostri amici medici, infermieri e professionisti della sanità: se pensate che questo provvedimento possa portare un beneficio rispetto al rischio di violenza che purtroppo oggi c'è nelle nostre strutture sanitarie, sappiate che purtroppo è una fiducia mal riposta, perché non è questo lo strumento da utilizzare. È inaccettabile - lo ha già detto il collega Scalfarotto, ma lo ribadisco anche io - questo continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, che meriterebbe ben altra riflessione e capacità di approfondimento, e non un decreto-legge. L'avete già fatto con il decreto-legge Caivano sulla violenza e sul disagio minorile. Avete fatto un disastro un disastro con quel decreto-legge: avete smantellato la giustizia minorile e avete riempito le carceri minorili di minori, mandando al collasso quei penitenziari senza risolvere minimamente il problema del disagio minorile. State ripetendo gli stessi errori continuamente, perché pensate che questo possa portare qualche voto in più. Per noi questa è cattiva politica, non è buona politica; è una politica che sbandiera, che cerca di produrre risultati che non verranno mai raggiunti semplicemente per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese. Noi ci asterremo perché si tratta di un provvedimento che cerca di dare una risposta, ma certamente non è questa la strada da seguire. Ci vorrebbero ben altre risorse, ben altra capacità e anche ben altra concezione della politica, che voi purtroppo non avete.

noi riteniamo che questo sia un provvedimento realmente importante, realmente efficace e che necessitava dello strumento della decretazione d'urgenza, perché l'approvazione di questo decreto-legge arriva in un momento in cui gli episodi di violenza contro il personale sanitario sono tristemente diventati una realtà quotidiana. Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute, solo nel 2023 sono state oltre 16.000 le segnalazioni complessive e le aggressioni a operatori sanitari sull'intero territorio nazionale, per un totale di circa 18.000 operatori coinvolti nelle aggressioni segnalate (la maggioranza delle vittime sono donne). Il fenomeno non è nuovo, considerato che per anni abbiamo assistito ad aggressioni al personale sanitario. È evidente che fin qui le azioni adottate e le normative approvate non sono state sufficienti ad arginare una piaga che - ricordiamolo rappresenta la prima motivazione di fuga all'estero di medici e infermieri del nostro Paese, accanto alla necessità di scegliere proposte economiche maggiormente gratificanti. La cronaca ha continuato a raccontare episodi di violenza incontrollata all'interno delle mura dei principali ospedali italiani.

In rete è stato diffuso un video di medici e infermieri barricati in una stanza per proteggersi dai parenti di una ragazza deceduta al Policlinico della città pugliese. Non c'è però solo Foggia, poiché le aggressioni si verificano in tutte le Regioni italiane. Questi eventi vanno analizzati nel complesso della loro gravità: è riduttivo pensare che si tratti esclusivamente di minaccia alla sicurezza fisica degli operatori, poiché incidono anche sul loro benessere psicologico, contribuendo al fenomeno del *burnout*, che colpisce già molte categorie professionali impegnate nel settore della cura e dell'assistenza, con ripercussioni sulla qualità del nostro Servizio sanitario nazionale. Per questo, al di là dell'inasprimento della pena edittale, si è ritenuto - e noi condividiamo pienamente questa scelta - che lo strumento più utile per cercare di combattere questo fenomeno inaccettabile, ovvero le aggressioni al personale sanitario, è quello di introdurre sempre l'arresto in flagranza del reato, anche differito. Non vogliamo più assistere a violenze nei confronti di donne e uomini del Servizio sanitario, e neanche alla distruzione di pronto soccorso e reparti. Queste misure si aggiungono ad altre già approvate lo scorso anno a scopo preventivo di deterrenza. Sono aumentate le pene per gli aggressori, è già prevista la procedibilità d'ufficio indipendentemente dalla denuncia di chi viene aggredito e sono stati potenziati i presìdi di polizia negli ospedali. I posti di polizia presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate nell'ultimo anno sono passati da 120 a 196 e il numero dei poliziotti negli ospedali è aumentato da 299 a 432. Con le novità introdotte dal decreto-legge in esame, il Governo Meloni vuole porre un freno agli episodi di violenza sociosanitaria. È un'altra risposta concreta del Governo a tutela di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, un'altra promessa mantenuta con chi ogni giorno si dedica con competenza e dedizione alla cura dei cittadini e non merita di essere oggetto di violenza. Dobbiamo essere consapevoli - e su questo mi auguro siamo tutti d'accordo - che quelli contro il personale sanitario non sono paragonabili ad altri reati di violenza o minaccia contro altri pubblici ufficiali. Chi lavora con grande fatica e sacrificio negli ambulatori e nei pronto soccorso si pone al servizio del cittadino nel momento più delicato della vita. Il fatto che vengano offesi, malmenati e devastati ambienti e strumenti essenziali è una cosa intollerabile. Vogliamo che nelle strutture sanitarie e sociosanitarie si lavori in sicurezza, ma sappiamo che accanto a questi doverosi e necessari interventi occorre uno sforzo ancora maggiore sul piano culturale. Per questo continueremo a promuovere, insieme alle categorie, campagne per sensibilizzare i cittadini e rinsaldare il rapporto di fiducia tra paziente e medico. Il diritto alla salute è un pilastro fondamentale della nostra società. Per garantire tale diritto, però, è necessario che chi lavora in questo settore possa operare in un ambiente sicuro e protetto. Accanto alle misure deterrenti e repressive che ho richiamato, è importante ricordare tutto ciò che in materia di prevenzione è stato proposto nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie ricostituito con decreto del Ministero della salute nel dicembre 2023, sta espletando un'attività di studio e approfondimento per ammodernare le raccomandazioni, predisporre *standard* minimi dei contenuti dei corsi di formazione rivolti a tutti gli operatori del settore sanitario e in previsione di adeguate campagne di comunicazione per sensibilizzare la popolazione, come strumento che riteniamo particolarmente efficace per ristabilire quel rapporto fiduciario cui ho poc'anzi accennato. L'intervento in discussione rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno che questo Governo sta mettendo in pratica per risollevare il nostro sistema sanitario nazionale. È uno sforzo che segue anni di carenza di programmazione e scarsa attenzione per il personale che opera nella sanità pubblica. Non esistono facili soluzioni, ma esiste un lavoro costante, fatto con competenza in un ambito delicato come quello del diritto alla salute, che sicuramente non ha bisogno di strumentalizzazioni, specie da chi in passato ha avuto la responsabilità della gestione della sanità pubblica e che solo adesso sembra aver preso consapevolezza delle gravi difficoltà in cui versa il nostro sistema sanitario. Peraltro, è per questo che trovo oggettivamente

È chiaro che questo è un provvedimento molto atteso dalla categoria degli operatori sanitari e che questo Governo ha avuto il coraggio, sotto forma di decreto, di intervenire con immediatezza su questo problema. che questa astensione voglia nascondere la volontà di dire: volevamo fare e non abbiamo fatto. Noi invece stiamo facendo e per questo dichiaro con convinzione il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.